del Regolamento, su misure di sostegno pubblico alla ricerca e al sistema universitario e problematiche connesse all'avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti,

che l'hanno incrementata e per le eccellenze dei singoli dipartimenti. Parte di queste ultime sono obbligatoriamente destinate all'assunzione di ricercatori, nonché ad un completo recupero dei tagli fatti negli ultimi anni alle università. Questi sono segnali che certamente vanno nella giusta

un finanziamento di 12 milioni di euro per l'educazione all'immagine e la formazione dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'incremento delle attività all'interno delle scuole di alta formazione per le professioni del cinema. Dall'analisi delle sue prime dichiarazioni non emerge quali siano le misure a sostegno degli enti di ricerca anche con riferimento alla particolare situazione contingente connessa allo schema di decreto legislativo per la semplificazione, attualmente in fase di esame parlamentare per l'acquisizione del prescritto parere. Le chiedo, pertanto, se e quali interventi siano previsti nella manovra

Le chiedo, inoltre, se sia previsto un sostegno per il reclutamento, considerata la centralità del capitale umano nel sistema ricerca. Signor Ministro, in Italia si spende in ricerca in misura minore rispetto alla media europea. Meno della metà della spesa è a carico del sistema pubblico e delle università; la rimanente quota è sostenuta dalle imprese, pur essendo il sistema industriale italiano formato largamente da piccolissime aziende, che sfortunatamente poco partecipano all'innovazione. Si registra, purtroppo, una scarsa collaborazione tra il sistema pubblico e quello delle imprese, soprattutto per quanto concerne l'applicazione pratica delle ricerche. Ministro, come si intenda mettere a confronto, si potrebbe dire a *network*, le differenti competenze pubbliche in tema di ricerca, che ora sono in capo a diversi Ministeri ed enti. Le chiediamo inoltre come si intenda rafforzare il sistema di relazioni tra gli enti di ricerca pubblici e il sistema universitario e come si intenda incentivare una strategia di lungo periodo per facilitare il dialogo tra il tessuto delle imprese e il vasto numero degli enti di ricerca italiani e delle università, al fine dell'utilizzazione delle ricerche da questi prodotti.

Considerato che il Trattato di Lisbona del 2000 e il trattato di Barcellona del 2002 fissano la soglia minima di finanziamento per ricerca e sviluppo al 3 per cento del PIL per il 2010,

negli ultimi anni si sta assistendo alla distruzione sistematica della ricerca e dell'università pubblica, si chiede al Ministro interrogato quali siano le reali misure volte al finanziamento della ricerca preannunciate subito dopo il Consiglio dei ministri. *(AP (NCD-UDC))*. Onorevole Ministro, per quanto concerne le misure relative a università e ricerca, lo scorso 29 giugno la Camera dei deputati, ad amplissima maggioranza, ha impegnato il Governo a rendere più eque dal punto di vista sociale e territoriale le politiche sull'università, a partire dal diritto allo studio e dalla ripartizione dei finanziamenti tra gli atenei. Il Governo, in particolare, si era impegnato ad assumere iniziative volte a garantire pari opportunità di accesso all'alta formazione universitaria, all'alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, attraverso un'effettiva implementazione del diritto allo studio, che valorizzi i talenti delle studentesse e degli studenti, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e i livelli europei ed internazionali. A tal proposito, la prossima legge di bilancio quali misure prevede in merito? Quali agevolazioni per i redditi medio bassi della popolazione per l'istruzione universitaria? In merito alla ricerca, si prevedono sgravi fiscali o agevolazioni di diversa natura, volti a favorire l'implementazione di tali attività nelle sedi universitarie? *(Misto-SI-SEL)*. Onorevole Ministro, nell'ambito delle misure di sostegno pubblico alla ricerca, questo Governo ha deciso di investire una consistente quantità di risorse nel progetto Human Technopole, affidandolo all'Istituto italiano di tecnologia proprio mentre si levano molteplici le lamentele per la carenza dei finanziamenti per università ed enti pubblici di ricerca, con particolare riguardo alla situazione di precarietà dei ricercatori. Tale modalità, che è ora oggetto di uno specifico affare assegnato in 7a e 12a Commissione qui in Senato, configura un cambio di rotta nella politica degli investimenti in ricerca, introducendo una modalità *top-down* che ha bypassato il sistema pubblico ed, in particolare, il sistema dei bandi competitivi per l'affidamento di questi progetti e, invece, si affida per decreto a fondazioni di diritto privato per la realizzazione degli stessi. Recenti inchieste giornalistiche, avallate dal *management* dell'Istituto italiano di tecnologia, hanno evidenziato come questa fondazione privata abbia messo da parte negli anni un tesoretto da 430 milioni di euro in un conto infruttifero della Banca d'Italia,

Lo stesso direttore scientifico della fondazione in questione, in una recente intervista televisiva, si è dichiarato addirittura favorevole ad usare questi fondi per scopi non direttamente riguardanti l'istituto

moltiplicando almeno di dieci volte il suo finanziamento. Quei colleghi non a caso hanno usato il verbo «salvare» perché di questo si tratta: si tratta di salvare un patrimonio che è destinato a svanire. Come lei sa, le procedure per l'assegnazione dei bandi PRIN si sono appena concluse: 92 milioni a disposizione per i prossimi tre anni dopo anni di finanziamento

almeno altri 500 milioni di euro per garantire continuativamente FIRB e PRIN decenti. Come ricordava il collega Bocchino, di questi 500 ben 430 milioni di euro sono disponibili pronta cassa su un conto infruttifero della Banca d'Italia. Si tratta di un accantonamento, che continua di anno in anno, di soldi pubblici destinati dallo Stato alla ricerca pubblica negli ultimi dieci anni. L'intestatario è l'Istituto italiano di tecnologia. Signor Ministro, le chiedo anch'io se è sua intenzione avvalersi di questa preziosissima liquidità per garantire la sopravvivenza, la sussistenza, l'esistenza della ricerca libera in questo Paese.

ci dicono che i sistemi universitari, per competere, hanno necessità di marciare di pari passo con la società e anzi, proprio da un sistema universitario avanzato dipende il futuro di un Paese, il suo posizionamento rispetto alle altre Nazioni. Alcuni dati statistici ci dicono che un anno di formazione in più può portare, in una nazione, all'uno per cento del PIL in più. In Italia il sistema universitario sembra muoversi tra un sistema formativo che non è più latino ma nemmeno pienamente americano, cioè caratterizzato dalla tensione verso la specializzazione, la produttività e la competitività. Si chiede di sapere se non sia opportuno sostenere il sistema universitario in maniera tale da garantire sempre più una maggiore specializzazione degli studenti da formare in tutte le branche, soprattutto in quelle scientifiche ma non solo, sia durante il percorso universitario sia in quello *post-*universitario, specializzazione che sarebbe opportuno rendere una tappa obbligata prima dell'accesso a qualsiasi professione. Le chiedo, inoltre, se non ritenga a tal fine necessario intervenire normativamente affinché ogni ateneo possa garantire tutte le specializzazioni, come pure se non ritiene necessario favorire il ricambio generazionale nel settore della ricerca universitaria al fine di immettere nel sistema energie più fresche e potenzialmente più protese alla crescita e alla

che «progressivamente abbandonasse la spesa storica a favore di criteri basati sulla premialità e sul costo *standard* per favorire una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'investimento pubblico nell'istruzione universitaria». Anche nel 2015 sono cresciute sia la quota premiale, dal 18 al 20 per cento, sia la percentuale della quota base assegnata in relazione al costo standard per studente, passata dal 20 al 25 per correggere l'assegnazione delle risorse, fino ad allora basata sulla spesa storica per cui chi più aveva ottenuto in passato più continuava a ricevere. Una volta a regime, l'intero fondo, dell'ammontare di circa 7 miliardi, verrà distribuito con criteri per il 70 per cento oggettivi (costi *standard*) e per il 30 per cento premiali, come nei Paesi più avanzati.

Sembra che il suddetto parere sia stato prontamente accolto dal Governo e qualcosa di simile temiamo succeda quando si andrà a definire il prossimo incremento della quota premiale, che a questo punto potrebbe limitarsi allo 0,5 per cento del FFO, ovvero il minimo per annualità previsto dalla legge n. 240 Quindi, signora Ministra, chiediamo: come giustifica il freno alla crescita dell'utilizzo di criteri oggettivi - cioè uguali per tutti - nell'assegnazione delle risorse, azione palesemente in contrasto con il principio legislativo dell'uguaglianza; se intenda effettivamente limitare al minimo l'incremento della quota premiale e quali azioni ritenga di intraprendere - lei, signora Ministra, della quale ci fidiamo - affinché le parole del *premier* Renzi - di cui non ci fidiamo - riguardo all'incremento di risorse per istruzione e ricerca non rimangano, ancora una volta, una promessa elettorale.

Come sappiamo, però, le precedenti manovre finanziarie hanno spesso contenuto misure insufficienti ed estemporanee, i cui principali effetti sono stati quelli di aumentare gli squilibri all'interno del sistema accademico e le disuguaglianze fra le sue componenti. Per quanto concerne le misure relative a università e ricerca, dovrebbe pesare la mozione del 29 giugno scorso, con cui il Parlamento, ad amplissima maggioranza, ha impegnato il Governo a rendere più eque dal punto di vista sociale e territoriale le politiche sull'università, a partire dal diritto allo studio e dalla ripartizione dei finanziamenti agli atenei. Infatti, il graduale impoverimento delle famiglie, il ceto medio in affanno e la disoccupazione crescente stanno restringendo gli spazi di accesso all'università

erogate le risorse del Fondo di finanziamento dell'università seguendo purtroppo i vecchi schemi e i vecchi criteri. Ora però i tempi dovrebbero essere maturi per capire se, su temi come diritto allo studio e reclutamento accademico, il Governo intenda dare respiro alle indicazioni del Parlamento o se voglia, invece, limitarsi a misure *spot*. Le proposte del Governo su diritto allo studio e reclutamento appaiono problematiche rispetto ai principi di equità sociale e territoriale nei punti di accesso e di autonomia dell'università italiana. Sicuramente sono insufficienti a risolvere i problemi. Come ha mostrato qualche giorno fa l'ultima indagine (ADI), che riunisce i dottorandi e i precari della ricerca, negli ultimi anni i posti di dottorato si sono quasi dimezzati, mentre rimane paurosamente alto il tasso di espulsione dei ricercatori non strutturati dall'università: per cento sarà costretto ad abbandonare la ricerca nei prossimi sei anni. Parliamo di migliaia e migliaia di persone, prevalentemente giovani. Soffre il sistema Paese e sono punti di PIL che evaporano. Per la somma di queste ragioni, signor Ministro, le chiedo se in occasione della prossima manovra di bilancio si riuscirà almeno a rendere strutturale il reclutamento aggiuntivo di ricercatori a tempo determinato e ad adottare, finalmente, alcuni correttivi sul dottorato di ricerca attraverso l'abolizione delle tasse.

una serie di aspetti che complessivamente ritengo possono essere riassunti come la visione del Governo sulle politiche e le modalità di finanziamento della ricerca universitaria e della ricerca svolta negli enti di ricerca pubblici italiani. toccati temi molto specifici, come il rapporto tra pubblico e privato, la semplificazione delle regole e delle procedure, il diritto allo studio e le misure più specificamente orientate alla cosiddetta ricerca di base. Ovviamente in una risposta di sintesi complessiva, di far riferimento a ciascuno dei punti toccati, ivi inclusi gli aspetti più di dettaglio, cui però chiaramente sento il dovere di rispondere,

specificare che per dare una risposta esaustiva si deve far riferimento puntuale a tutte le misure che nel corso di questo triennio il Governo ha dedicato all'università e alla ricerca e che ha indirizzato a due fondamentali capitoli: il finanziamento e la valorizzazione dei progetti e delle attività di ricerca e il finanziamento e la valorizzazione del capitale umano. Sa molto bene la senatrice Cattaneo, che è un'autorevole esponente del mondo accademico al di fuori di quest'Aula (e lo è ovviamente anche qui), che tutto ciò che è finanziamento del capitale umano è sostanzialmente finanziamento della ricerca di base, perché essa, sia pur in forma non dedicata al singolo progetto, viene svolta, nei laboratori, nelle biblioteche, nei settori umanistici e in quelli scientifici, dalle persone, in particolare dalle giovani persone (dal dottorato, al *postdoc*, ai ricercatori) che sviluppano il progresso del pensiero scientifico. Citerò quindi anche le misure che riguardano la valorizzazione del capitale umano, ritenendo che esse siano parte integrante delle misure che il Governo dedica alla ricerca di base. Partiamo però puntualmente dalle ultime due leggi di stabilità, che hanno segnato un' inversione di tendenza netta, chiara, misurabile e quantificabile rispetto a quanto avvenuto nel precedente decennio. Il Fondo di finanziamento ordinario, che lo scorso anno era stabilizzato a 6,9 miliardi, nel 2018 salirà a 7,323 miliardi, una cifra che non era

però solo di un problema di quantità complessiva, è un problema e un tema di differente assegnazione di questi fondi, con una valorizzazione della premialità e con un obiettivo di innalzamento della qualità della ricerca scientifica e della didattica universitaria, che - non dimentichiamolo - sono due lati di una stessa medaglia. A questo riguardo vorrei ricordare che, sempre nella legge di stabilità 2016, sono stati aggiunti 25 milioni di euro in quota premiale

i numeri dei giovani che potranno trovare collocazione nelle nostre università, a partire dai dottorati di ricerca, avanzando nella scala di carriera e di evoluzione professionale, siano l'effettivo motore del progresso scientifico, e quindi il primo fondamentale strumento di finanziamento della ricerca di base. Questo non è comparabile con altri sistemi, come sanno bene gli onorevoli senatori che si sono pronunciati sul punto, perché è chiaro che in un sistema anglosassone, un sistema angloamericano, in cui il sistema universitario non ha finanziamento pubblico finalizzato all'assunzione e al reclutamento, quel capitolo non è finanza pubblica per la ricerca di base. Quindi, i sistemi di quel tipo finanziano fondamentalmente a progetto i migliori atenei, i migliori dipartimenti, i migliori noi facciamo questo, ma in misura diversa e con una scalarità che non è paragonabile. Vengo alla descrizione sintetica delle misure specifiche su questo punto, che mi preme molto. Voglio citare dal 2015 ad oggi l'adozione del piano straordinario di assunzioni per i professori di prima fascia,

ricercatore di tipo A; l'assunzione di un piano - lo dicemmo lo scorso anno e lo ribadisco con dati oggettivi e quantificabili quest'anno - non straordinario, ma che diventa strutturale e permanente, di 1.027 ricercatori lo scorso anno per l'università e la quota restante per gli enti di ricerca) e che quest'anno sarà possibile continuare. Infatti, grazie a un'altra misura che ha una finalità aggiuntiva rispetto all'assunzione diretta, ma le cui risorse vanno anche all'assunzione diretta, e cioè quella quota destinata alla valorizzazione dei dipartimenti dipartimenti eccellenti, ovvero quelli che dimostrano una qualità di ricerca valutata sulla base della nuova VQR al di sopra di un certo *standard*,

è un unico processo che si svolge in luoghi diversi nel nostro Paese, ma che deve avere analoghe, commisurate e coerenti risposte. per quanto riguarda trasferimento tecnologico e contatto maggiore con il mondo dell'impresa, e comunque con il processo produttivo, richiamo un'altra misura importantissima, che è il capitolo relativo a *enabling factors*, competenze e formazione del Piano industria 4.0, che è il grande progetto progetto avviato, con il coordinamento del ministro Calenda, di cui il nostro Ministero sarà portatore e coordinatore per una serie di azioni, quali la valorizzazione e il potenziamento degli istituti tecnici superiori, che sono quell'istruzione terziaria che non è non è estranea ai ragionamenti che stiamo facendo, e in cui il nostro Paese ha gravi lacune di qualità e di quantità. Cito, poi, naturalmente i c*ompetence center*, che diventano laboratori attivi e sono la novità anche strutturale per collegare meglio e, come lei richiama,

al merito abbinato al bisogno, cioè alla valorizzazione delle qualità (articolo 34 della nostra Costituzione) in abbinamento a condizioni non sempre agiate delle famiglie di partenza: ricordo che questa misura consentirà a circa 400 borsisti, ritenuti altamente meritevoli sulla base dei *curricula* ricavati dalle scuole superiori, di avere un accompagnamento completo nel percorso universitario, con borse di studio che non coprano soltanto la parte dell'iscrizione e della tassa universitaria, ma che accompagnino tutto il percorso, con 15.000 euro circa di copertura: è una misura direi assolutamente eccezionale per il nostro Paese.

all'attività scientifica dei nostri atenei, ma anche dei nostri enti di ricerca. Ricordo tutte le misure che sono già state inserite nel Piano nazionale (che, lo ricordo, destina al capitale umano 411 milioni di euro), di cui il progetto Dottorati innovativi è il segmento altamente qualificante. Non cito altri progetti più specifici, che rientrano sempre in misure di finanziamento della ricerca di base, fatto salvo uno che è molto importante e riguarda i 246 milioni di euro previsti per l'accompagnamento e il cofinanziamento dei ricercatori che siano vincitori di questa è una misura del tutto innovativa, che consentirà non solo ai vincitori che vorranno restare in Italia, se sono italiani, ma soprattutto costituirà un un elemento di forte attrattività per coloro che si trovano all'estero. la senatrice Cattaneo e il senatore Bocchino e che riguarda l'Istituto italiano di tecnologia e il presunto - fonti di stampa, ma a noi non risulta - tesoretto, così come è stato definito. Chiaramente l'Istituto italiano di tecnologia è responsabile, con trasparenza, del proprio bilancio.

GIORGI *(PD)*. Signor Ministro, sono abbastanza soddisfatta della sua risposta. Ritengo tuttavia che ci sia ancora del lavoro da fare e credo che ce ne faremo carico come Parlamento. Infatti, rispetto alla necessità di interventi importanti in questo mondo, indubbiamente ancora si mantiene, secondo la mia opinione, un certo squilibrio nelle misure in favore delle università rispetto agli enti pubblici di ricerca, anche se concordo sulla sua impostazione secondo cui la ricerca è un tutt'uno. Proprio per questo credo che, sulle risorse umane, si debba fare uno sforzo ulteriore, anche per questo settore che assorbe moltissimo dell'intervento pubblico nel settore della ricerca. questione di cui parlava, anch'io le avevo posto la domanda relativamente al diritto allo studio e mi sembra molto interessante la risposta che viene data quest'anno da questa legge di bilancio.

del nostro Paese (la Germania, ad esempio, ha una percentuale doppia). Siamo convinti che debbano essere prese iniziative durature, se il Piano quell'apporto che noi vogliamo per favorire il coinvolgimento delle imprese nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo, e che debba essere comunque agevolata in ogni modo una maggiore interazione con il sistema della ricerca pubblica. Presidente, ringrazio la Ministra per i dati che ha snocciolato a profusione (lei è molto brava a fare questo); rimane comunque una preoccupazione. La Ministra ci viene a parlare di una legge di stabilità come se fosse stata già approvata,

la ricerca ha bisogno di investimenti strutturali e, quindi, avrebbe bisogno anche di misure che vadano oltre i piani triennali, piani settennali, così come doveva essere l'iniziativa dei famosi 500 professori. Ci chiediamo quale professore verrà in Italia senza la certezza di avere finanziamenti strutturali alla ricerca.

della ricerca e aumentare la quantità degli studenti universitari. Effettivamente è necessario guardare anche ai meritevoli, che magari si trovano in situazioni difficili dal punto di vista economico: anche questi hanno diritto allo studio. Per quanto riguarda la ricerca, effettivamente sono state potenziate le risorse rispetto alle finanziarie precedenti; tuttavia riteniamo che, affinché l'Italia resti un Paese competitivo a livello internazionale, si debba investire molto in questo settore. Naturalmente lei ha fatto riferimento anche al lavoro che dovrà essere svolto a livello parlamentare durante l'*iter* di approvazione

non ha alcun senso e contribuisce a esacerbare ancora di più le differenze. Da questo punto di vista avevo suggerito l'uso del famoso tesoretto, proprio per mettere in sicurezza il sistema con interventi strutturali.

di questi soldi, che esistono, sono lì e sono ben documentati.

accantonati appartengono alla missione 17 del MEF, denominata «Ricerca e innovazione», programma 15 «Ricerca di base e applicata». Quello che le sto chiedendo non è una concessione a favore della ricerca libera, ma piuttosto che fondi iscritti al bilancio dello Stato, dedicati alla ricerca pubblica, siano finalmente impiegati in quella direzione, siano quindi liberati insieme alle idee di tutti gli studiosi d'Italia. auguro veramente che lei possa farsi alfiere di questa richiesta nel prossimo *iter* parlamentare, perché sarebbe un segnale importantissimo per tutti gli studiosi di tutti gli ambiti disciplinari d'Italia.

la invitiamo a fare di più (la lode non gliela diamo, visto che parliamo di università). Le chiediamo di favorire il *turnover* con uno

sempre, infatti, chi è giovane è bravo, e non sempre chi è anziano è demotivato. Le ricordo che una collega, Rita Levi Montalcini ha avuto il premio Nobel a settantaquattro anni, quindi era un'anziana brava. Di conseguenza, noi vogliamo che gli anziani che riescono a fare scuola rimangano e che quelli demotivati (grosso modo, quelli della mia età), che non hanno più alcun tipo di motivazione e non fanno più ricerca,

Penso che, nel momento in cui i rettori e la CRUI stanno lanciando un grido d'allarme nei confronti del Governo e di chi amministra questo Stato, bisogna tenerlo in considerazione,

signora Ministra, sono parzialmente soddisfatto per una ragione: la necessità di capire che cosa succede di quel 93 per cento di ricercatori che nei prossimi sei anni saranno espulsi dall'università, o meglio dal circuito della ricerca. Sono convinto che lo zelo e l'attenzione che la Ministra mette nell'applicarsi al ruolo che svolge

l'attuazione della riforma della scuola comporta maggiori oneri in termini di qualità dei servizi offerti all'utenza e quindi richiede un'implementazione di dotazione di personale docente e ATA. È evidente che una riforma profonda e strutturale, quale quella approvata lo scorso anno, necessita tempo per esplicare i suoi effetti a regime. Sono però innegabili i problemi di gestione derivanti dalla mobilità straordinaria che ha coinvolto 200.000 lavoratori e le criticità, relative a procedure, tempistiche e contenziosi in gran parte eredità di un precariato stratificato in troppi anni. L'importante operazione del concorso, un punto qualitativamente rilevante della riforma, ha incontrato ostacoli in grado di rallentarne le procedure. Pur con le dovute differenze tra Regioni - personalmente ho presente la situazione del Piemonte - nelle prossime settimane nelle scuole si stabilizzerà la situazione dei docenti con il reclutamento dalle GAE

dalle molte reggenze e dall'attuale situazione del personale amministrativo, in particolare in relazione ai direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Certa e consapevole del fatto che queste difficoltà non devono ledere l'efficacia della riforma, ma altrettanto consapevoli che è indifferibile il superamento delle stesse per dare una risposta efficace al mondo della scuola, le chiedo, signora Ministra, di conoscere quali sono i motivi che hanno portato alla criticità dell'avvio dell'anno scolastico e che rischiano di ostacolare il regolare svolgimento delle lezioni con una conseguente riduzione dell'offerta formativa. Le chiedo altresì di sapere in che modo la gestione della mobilità ha influito su questa situazione quali notizie ci può dare sull'emanando corso-concorso dei dirigenti scolastici e dei DSGA al fine di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico. ha facoltà. PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, vorrei porre alla sua attenzione un aspetto specifico legato al reclutamento dei docenti, questione che sta creando molte difficoltà al corretto inizio dell'anno scolastico. Mi riferisco ai 45.000 docenti delle liste graduatorie ad esaurimento (GAE) che hanno deciso di non aderire al piano di assunzioni previsto dalla buona scuola, a causa della cosiddetta disponibilità nazionale, che imponeva di accettare qualunque sede di lavoro proposta, e dell'impossibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria vicino casa nell'ipotesi di trasferimento in una sede lontana, con rischio di cancellazione dalle graduatorie in caso di rifiuto. Queste ragioni sono state successivamente accolte nella legge n. 42 del 29 marzo di quest'anno, purtroppo però quando i termini per aderire al piano delle assunzioni erano già scaduti, con danno evidente per i docenti della graduatoria in questione. pertanto, se sia previsto un futuro e prossimo piano di svuotamento delle liste delle graduatorie ad esaurimento e una qualche forma di tutela o graduatoria preferenziale

l'anno scolastico, ancor più del precedente, ha evidenziato tutti gli aspetti negativi della buona scuola ed è iniziato con moltissimi problemi, a cominciare dai circa 60.000 bambini senza sostegno per mancanza di nomina dell'insegnante. Fino alla metà di ottobre sono rimaste 10.500 cattedre vuote e c'è una sostanziale mancanza di chiarezza sulle assunzioni e sugli aventi diritto. Non possiamo continuare a ignorare docenti precari abilitati con un serio e costoso percorso SSIS e vincitori di concorso che hanno deciso di non partecipare al piano di assunzioni previsto dalla legge non volendo affidare il proprio destino al misterioso algoritmo che li avrebbe costretti a trasferirsi lontani con uno stipendio medio di 1.300 euro. Le scelte che avete voluto fare per risolvere la differenza quantitativa del precariato tra Nord e Sud, inventando le assunzioni sul potenziamento in classi di concorso diverse e senza rispondenza alle cattedre vacanti, si sono rivelate fallimentari. Ancor più si è rivelato ingiusto e dannoso il successivo emendamento

ci sono lavoratori fuori dal mondo della scuola. Signora Ministra, gli insegnanti precari storici delle GAE con più di trentasei mesi di servizio vorrebbero sapere se esiste la concreta possibilità di vedere riconosciuto il diritto all'assunzione diretta... giuridica, senza dover ricorrere alle vie legali. Saranno trasformate le cattedre attualmente in organico di fatto Sono previsti corsi per l'abilitazione di chi ha lavorato per anni nelle scuole? Per le insegnanti della scuola dell'infanzia, che non hanno visto riconosciuti fino ad oggi i propri diritti? PRESIDENTE. Deve concludere, altrimenti toglie la parola agli altri.

onorevole Ministro, le operazioni relative ai trasferimenti dei docenti ed il concorso per le nuove assunzioni hanno avuto tempistiche molto più lunghe del previsto. Allo stato attuale, risultano pendenti molti ricorsi, il cui esito potrebbe alterare le graduatorie utilizzate per la copertura dei posti disponibili, innescando un processo di spostamenti di cattedra che andrebbe a minare la continuità didattica. In alcune aree del Nord molti posti risultano tuttora non coperti, anche dopo le chiamate da parte degli uffici scolastici provinciali, perché le relative graduatorie sono esaurite. La copertura dei posti sarà possibile solo ad anno scolastico inoltrato e ricorrendo alle graduatorie di istituto. Risultano inoltre scoperti anche molti posti di dirigente scolastico per i quali si è reso necessario ricorrere all'assegnazione di molti incarichi di reggenza. Si chiede di sapere se tale situazione era stata presa in considerazione dal Dicastero da lei rappresentato e quali iniziative si intendano assumere, soprattutto in relazione ai ricorsi pendenti, per consentire il regolare proseguimento del corrente anno scolastico, evitando in futuro analoga situazione. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, si chiede di conoscere quali misure si intendano adottare considerate le vacanze di posti in organico e se se siano ipotizzabili iniziative per eliminare il contenzioso in essere. quest'anno le scuole stanno sperimentando più che mai la mancanza di docenti, sia su posti comuni che su posti di sostegno, ricorrendo alle supplenze, peraltro fino agli aventi diritto. Stiamo assistendo ad un cambio continuo di docenti, prima nominati con la più che discutibile chiamata diretta e poi revocati d'ufficio dall'incarico sopraggiunto per un nuovo docente.

PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Ministra, con bando del luglio 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici: ben 2.386 i posti complessivi, di cui 224 per la Campania. Bene, 50 docenti campani non hanno superato la prova preselettiva. Tuttavia, il TAR Campania, accogliendone l'istanza, li ha ammessi alle prove successive, sia scritte che orali, che sono state superate dagli stessi con esito positivo. Con successivo provvedimento dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, tali docenti sono stati però esclusi, nonostante la già citata decisione giurisdizionale. A sostanziale fondamento di questa interrogazione e di questa controversa vicenda, rilevo una palese disparità di trattamento in quanto, per situazioni identiche, i ricorrenti di altre Regioni sono stati inseriti nella graduatoria di merito. Ciò premesso, chiedo a lei, signora Ministra, se e come ritenga opportuno intervenire per definire la situazione dei succitati docenti

BARANI *(AL-A)*. Signora Ministra, ogni avvio di anno scolastico è interessato da problemi che riguardano l'assegnazione delle cattedre ai docenti, come pure quelli che riguardano l'assegnazione dei posti al personale ATA. In realtà, da un po' di tempo siamo abituati a vedere un mese di settembre caratterizzato dalle supplenze e mai da docenti fissi, che poi accompagneranno gli alunni per tutto l'anno scolastico. Poiché questo stato di disagio e di diffusa confusione sembra essere diventata una costante dell'inizio di ogni anno scolastico, si chiede, a prescindere da ogni valutazione sulla riforma della scuola, sul tema dei pensionamenti, sugli esiti dei concorsi e delle assunzioni a tempo determinato e del ruolo del personale ATA, se non ritenga opportuno anticipare la valutazione di tali problemi ad un tempo poco poco a ridosso dalla fine del precedente anno scolastico, così da affrontare tutte le varie problematiche del reclutamento e assegnazione dei docenti durante il periodo estivo, potendo esaminare ricorsi, impugnazioni e quant'altro in tempo utile

docenti, lo svecchiamento, onde consentire di immettere nel sistema dell'insegnamento energie più fresche e di attribuire specifiche competenze, in questo senso, agli uffici scolastici provinciali

Signor Ministro, la ringrazio per essere qui di persona. Venendo al dunque, nelle scuole italiane mancano gli insegnanti di sostegno, figure spesso dimenticate ma indispensabili perché tanti dei nostri ragazzi in difficoltà riescano comunque a prepararsi e ad affrontare la vita. Per esempio a Napoli, all'Istituto comprensivo 73 «Michelangelo Ilioneo», dove, a fronte di 20 ragazzi bisognosi di sostegno e di ben 14 sentenze del TAR che riconoscono complessivamente 441 ore di copertura, sono assegnati solo 16 docenti di sostegno contro i 24 che sarebbero necessari a sostenere solo i ragazzi per cui le famiglie hanno ottenuto le sentenze di assegnazione. Ci domandiamo se gli altri sei ragazzi, quindi, siano poveri. Mi preme chiedere al Ministro quando sarà disponibile l'organico previsto dalla normativa, non solo per la scuola «Ilioneo»,

Signora Presidente, qui veniamo al dunque, perché la scuola è l'esempio del fallimento del Governo Renzi, dal momento che la prima volta che è venuto in quest'Aula, seduto due posti più in là rispetto al Ministro, il presidente Renzi ci aveva detto che la scuola sarebbe stata la priorità di questo Governo. Come lo scorso anno, signor Ministro, le scuole hanno riaperto senza decine di migliaia di insegnanti titolari, solo in parte sostituiti da figure provvisorie con docenti che in molte classi sono cambiati rispetto all'anno precedente, a tutto discapito della continuità didattica, e con un istituto su sei senza dirigente scolastico. Se per tanti insegnanti del Sud, dove storicamente un elevato numero di persone punta su questo tipo di impiego, finora il trasferimento in un'altra Regione era comunque una scelta sofferta e non un obbligo, dopo la legge n. 107 del 2015, meglio nota come la buona scuola - ahimè - il trasferimento è diventato un'imposizione. I neoimmessi in ruolo nella fase C, infatti, hanno dovuto esprimere tante preferenze quante sono le Province, scegliendole magari in base al parente che poteva ospitarli per poter risparmiare. Conseguentemente, non si verificano più solo trasferimenti dal Sud al Nord ma anche spostamenti fuori dalla propria Regione per migliaia di docenti del Centro-Nord dove ci sono più posti da coprire che insegnanti a cui assegnarli. Questa disaffezione nella scelta delle sedi al Nord è generata principalmente dal costo della vita che, a parità di emolumenti, al Nord è superiore del 30 per cento. Stiamo ricevendo, anche sulle nostre *mail* istituzionali, migliaia di proteste da parte di docenti, che si ritrovano letteralmente deportati da una parte all'altra della Penisola, con familiari e figli anche piccoli al seguito o che sono costretti a lasciare nelle zone d'origine, con il rischio di lavorare in perdita, vista l'esiguità dello stipendio degli insegnanti italiani. Quindi, signor Ministro, le chiediamo se alla luce della situazione sopra descritta, che sicuramente è ben nota al Ministro, il Governo non stia seriamente valutando la possibilità di modificare l'attuale meccanismo di reclutamento degli insegnanti, attraverso concorsi nazionali a gestione regionale, ai fini di risolvere le situazioni negative sopra descritte, nelle quali perdono tutti i soggetti in gioco, a danno della qualità dell'insegnamento nel nostro Paese. giungono dalla periferia del Paese notizie poco rassicuranti sulla scuola: le lezioni si svolgono a singhiozzo, le classi vengono continuamente smembrate e un alunno disabile su tre è ancora senza insegnante specializzato o in procinto di cambiarlo. Se secondo i dati in possesso del Ministero così non è, saremo felici di essere smentiti da lei, ministro Giannini, che ci sta mettendo la faccia, come oggi usa dirsi. La situazione è quella di avere un professore di ruolo su sei, mentre decine di migliaia di docenti di ruolo ancora devono essere utilizzati e assegnati agli istituti; 100.000 sono gli insegnanti precari, di cui 40.000 di sostegno, che attendono la nomina annuale

del potenziamento. Non è il collasso - per carità - non ci piace fare facile demagogia, ma la precarietà si percepisce e il *sentiment* del Paese ne è pervaso. Si spera di poter sopperire alla *vacatio* con i vincitori del concorso, ma le graduatorie di merito vanno a rilento e i vincitori sono comunque pochi in tutta Italia, a causa dell'altissima percentuale di bocciature. Siamo al paradosso: prima c'erano i tagli e non si poteva assumere. Quest'anno lo Stato ha messo le risorse, ma l'organico di fatto non c'è. Quali sono, quindi, le misure urgenti che si stanno ponendo in essere per arginare questa situazione? Tutto l'anno scolastico si svolgerà

corrisponde un'omogeneità maggiore rispetto alla complessità dei precedenti quesiti, riguardanti l'università e la ricerca, in quanto sono concentrati essenzialmente sui problemi e i temi riguardanti il personale della scuola. dunque una legittima e, dal mio punto di vista, anche doverosa indicazione di risposta a tutte le singole questioni. Voglio ricordare che la legge n. ha mirato a introdurre importanti e cruciali innovazioni, che riguardano anche e soprattutto gli studenti, che sono il centro dell'attività didattica della scuola. Probabilmente, signora Presidente, avremo un'altra occasione per discuterne. caso mi concentrerò su tre o quattro blocchi di domande, cercando anche di far riferimento ai singoli quesiti. Mi riferisco alla complessità o alle criticità che hanno riguardato l'avvio dell'anno scolastico in relazione a due fondamentali processi, che hanno carattere di straordinarietà e che, francamente, mi permetto di valutare come la risposta (con questa legge) al fallimento sulla scuola di una discreta quantità di Governi che ci hanno preceduto. si è concentrata su un'azione fondamentale: un piano assunzionale che lo scorso anno ha portato all'immissione di 120.000 docenti, di cui 47.000 per potenziamento. Potenziamento significa dare più insegnanti alle scuole, qualificarne le specializzazioni e quindi avere una ricaduta importante sulla didattica e sull'offerta formativa delle scuole medesime; significa anche assegnare cosa che non era stata fatta nei precedenti decenni - un diritto alla stabilità di vita e di posizione nello Stato, ai sensi della Costituzione italiana. Questi numeri imponenti si sono poi abbinati a un altro processo, ben noto agli interroganti, indicato dalla legge e introdotto nella legge dal percorso parlamentare, come è ovvio e giusto che avvenga, cioè il piano straordinario di mobilità dei docenti, che ha riguardato 207.000 posizioni che si sono potute rimettere in discussione nella loro collocazione collocazione e nella destinazione finale. L'intreccio di questi due fattori, ha creato una maggiore complessità in questo anno scolastico nell'assegnazione dei ruoli e delle cattedre.

Le assegnazioni e le situazioni critiche che in queste recenti settimane sono state collegate alle assegnazioni provvisorie, all'intreccio di questo piano straordinario di mobilità e del contratto di mobilità, che ha cambiato il sistema dei trasferimenti rendendoli anche interprovinciali, all'introduzione della novità rilevante dei cosiddetti ambiti rispetto a quanto era prima, cioè la semplice elencazione per punteggio e per graduatoria. Tutto questo ha creato un sistema che in questi giorni si sta aggiustando, naturalmente con un fenomeno che in qualche caso è irrisolvibile. Cito il caso delle cattedre di matematica, evocato da ultimo dal senatore Liuzzi, che in qualche frangente sono anche rimaste scoperte nella messa a concorso della stessa classe di concorso. Purtroppo questo lo si risolve soltanto lavorando dal basso e facendo sì che aumentino gli iscritti nelle facoltà scientifiche, in particolare di matematica, e che i laureati in tale materia possano avere un avvio regolare della loro carriera di insegnante, con una procedura regolare che non sia il il decennio o il ventennio di precariato, ma un concorso nazionale che possa dare giovani preparati e motivati alla scuola italiana. Il tema fondamentale che non era stato ancora risolto e che in questa legge di stabilità avrà un'opportunità di essere risolto, perché è il convitato di pietra di tutti questi temi che abbiamo discusso (e che in altre occasioni sono stati commentati con i dati precisi che vi ho riferito e che continuerò nel dettaglio a citare), è quello della discrasia tra un organico di fatto e uno di diritto. Questo è il vero tema della scuola ed è quello che nel corso degli anni ha creato le complessità di base nell'assegnazione dell'organico. Ricordo che per la prima volta in questa legge di stabilità nel Fondo unico che riguarda la pubblica amministrazione è stata destinata una somma precisa alla risoluzione di questo problema. Sarà quindi una Sarà quindi una grande opportunità, che non riguarda solo il Governo, ma il confronto tra l'Esecutivo e le forze sindacali, affinché questi fondi possano definitivamente essere assegnati alla trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto. Insieme Insieme alle assunzioni e al concorso in atto, questo sarà il vero motore di una stabilizzazione del personale docente che, mi sembra di capire, è il tema fondamentale che loro sollevano alla mia attenzione.

accedere al mondo della scuola. Non è un concorso straordinario, è stato straordinario per numeri (63.700 cattedre, come ricorderete, messe a concorso), ma diventerà il meccanismo che, con cadenza triennale, con gestione nazionale ma su base regionale - senatore Centinaio, rispondo anche alla sua sollecitazione potrà consentire a chi si laurea di entrare nel mondo della scuola attraverso la porta principale, riformando anche - c'è una delega specifica che riguarda questo capitolo, come ricorderete - il sistema di formazione iniziale dei docenti, e quindi l'accesso al concorso: altro obiettivo della legge Il concorso in atto è completato per il 55 per cento delle procedure che erano state attivate; ha riguardato ad oggi 21.640 posti per il triennio 2016-2018. Ricordo ancora una volta che tutti coloro che hanno partecipato da vincitori a questo concorso saranno assunti nel corso del triennio, come prevede la legge e com'è garanzia necessaria e doverosa nei confronti dei partecipanti. Per quanto riguarda l'altro tema, che diversi senatori hanno sollevato, e cioè cosa succede alle graduatorie ad esaurimento, ricordo che sono state un obiettivo specifico di questo Governo perché ritenute, e non solo da questo Governo, un'anomalia del sistema. È insito insito nella definizione stessa di graduatoria ad esaurimento l'idea che si accumulino centinaia di migliaia di persone con una prospettiva di stabilità impossibile e che queste persone debbano aspettare un altrettanto utopistico orizzonte di assunzione. Con le operazioni massicce

legge n. 107 e il riferimento che essa fa al testo unico sull'istruzione per quanto concerne questo capitolo, che è l'articolo 399, comma 1. Questo significa che, fino al momento in cui

dalla senatrice Ferrara, sono stati un obiettivo fondamentale nel potenziamento quantitativo e nella loro valorizzazione qualitativa. È il primo concorso che introduce, non dimentichiamolo, classi specifiche per il sostegno; sono aumentati complessivamente del cinque per nel nostro Paese) e credo che non esista altro Paese europeo che abbia questi numeri per questa importantissima categoria di personale qualificato del mondo della scuola. Abbiamo una delega che riguarda la disabilità

Mi si chiede quando e come sarà potenziata questa categoria professionale del mondo della scuola. Ricordo che è stata garantita e autorizzata l'immissione in ruolo di 285 nuove figure di dirigente scolastico. Ricordo che, a questo punto, è il Ministero dell'istruzione, dopo una prima fase in la gestione alla Scuola della pubblica amministrazione, che sarà gestore in prima persona del concorso: ciò consentirà di limitare le reggenze in maniera drastica (oggi sono 1.400 a fronte di un totale di 7.200 dirigenti scolastici), calcolo molto preciso, alle sole 335 scuole sottodimensionate. Quindi, nell'arco di un anno e mezzo, il fenomeno della reggenza avrà una drastica riduzione, determinata da questo fatto. Sempre sui dirigenti, c'è una domanda puntuale del senatore Romano che riguarda il caso Campania: ricordo che la legge, ai commi 87-91, ha inteso risolvere uniformemente, a livello nazionale, sia le questioni di portata generale, come l'annullamento della procedura, che è stata affrontata senza un'indicazione geografica, sia quelle che si sono poi prolungate nel tempo e che vedevano diverse situazioni di gestione nelle differenti Regioni. Tra la platea dei destinatari non rientra la fattispecie dei ricorrenti della Campania, per i quali si dovrà naturalmente attendere l'esito definitivo dei ricorsi, sulla base del quale vedremo poi quali misure adottare.

È un dato che, in questa circostanza, è emerso con maggiore forza per i numeri che ho citato, riferiti al piano assunzionale, alla mobilità straordinaria e al concorso in atto.

Il meccanismo concorsuale che ho indicato, con la modalità che citavo, sarà, nella prospettiva, una risposta molto precisa anche a questo tipo di fenomeno. Credo comunque che non sia corretto immaginare, in un Paese unico, unitario e sostanzialmente unito nella sua identità culturale, linguistica e nel suo assetto istituzionale, che sia un male assoluto essere oggetto di trasferimento, per una fase della vita e della propria carriera nel settore pubblico, che sia la scuola o qualcos'altro, in un'altra parte del Paese. Quello che è importante è che questo diventi un processo governato e governabile e che non sia frutto di di un'obbligatorietà. Non lo è stato con la legge n. 107, lo voglio ricordare, perché il piano assunzionale ha prospettato l'opzione di trasformare, per chi aveva un ruolo precario, quel posto in un ruolo stabile e negli anni precedenti lo spostamento avveniva, sì, ma per fare supplenze, sempre con la stessa traiettoria: dal Sud verso il Nord. Credo che anche in questo senso sia stato fatto un gigantesco

poco generose - lo dico qui - le accuse generalizzate che vengono lanciate. Vi sono sicuramente situazioni particolari e criticità. La collega Ferrara ne aveva poste alcune rispetto a situazioni di effettiva difficoltà che vengono a definirsi. Comunque, molte di esse sono in via di soluzione, come il Ministro diceva.

Il vero motore, Ministro, era proprio quello di stanziare delle somme precise per il problema dell'organico di fatto e dell'organico di diritto e la legge di stabilità c'è stata anche l'anno scorso, si poteva prevedere lì. Comunque, per quanto riguarda il numero alto di insegnanti di sostegno, dovremmo intanto capire come mai in Italia assegniamo al sostegno una serie di bambini che invece dovrebbero essere trattati in modo diverso, perché ancora non definiamo con chiarezza cosa sia un disabile.

la realtà nelle scuole è tutt'altra. Le scuole - e non lo avremmo mai detto - sono nel totale caos, così come negli anni precedenti, in perfetta continuità

la quale lei è stata così omissiva: capiamo che assistere al fallimento della buona scuola dopo un anno dalla sua approvazione è un duro colpo per il Governo.

della materia: ogni riforma della scuola è sempre stata contestata, dalla Gentile, alla Gelmini, alla Moratti, alla sua. In attesa che anche i tribunali amministrativi entrino a gamba tesa sul personale (e quelli vanno ascoltati) e in attesa di fare una scuola sotto casa di ogni dipendente e di ogni insegnante, cosa che non è possibile, noi riteniamo che lei stia facendo un buon lavoro. La invitiamo ad accelerare il *turnover*, lo svecchiamento, perché c'è bisogno di introdurre giovani più preparati nella scuola,

solerzia e l'attenzione con cui ha risposto ai problemi della nostra scuola. Mi ritengo però parzialmente soddisfatto perché mi permetto di ribadire che la situazione di fatto è che nelle scuole italiane mancano gli insegnanti di sostegno. Quando sarà disponibile l'organico previsto dalla normativa, non solo per scuole di Napoli ma per tutte le scuole d'Italia, per tutti i ragazzi d'Italia e per tutti quelli che non possono permettersi una sentenza del TAR? Signor Ministro, la buona scuola è un disastro, le scuole belle invocate dal senatore Barani altrettanto, visto che quasi settimanalmente abbiamo un soffitto che crolla o una scuola messa in condizioni pessime, e soprattutto abbiamo i genitori che quasi devono portare anche la carta igienica per i propri figli. Ma ricordiamo alcune cose. Signor Ministro, la transumanza da Sud a Nord c'è sempre stata, noi vogliamo evitare che ci sia anche la transumanza da Est a Ovest o da Ovest a Est. Il nostro obiettivo e il nostro sogno è che un insegnante possa insegnare non sotto casa, ma almeno nella propria Provincia, come accade a qualcuno che abita a Firenze ed insegna sotto casa. Sapevamo che la mobilità straordinaria prevista questa estate avrebbe modificato pesantemente la situazione, quindi, secondo noi, non aveva senso varare un concorso prima della mobilità. Poi lei, signor Ministro, continua a darci dei numeri stratosferici. Il problema di fatto è che i numeri non coprono nemmeno il *turnover*. Quest'anno, l'anno scolastico è iniziato con 40.000 insegnanti di sostegno in meno: se questa è la buona scuola, se queste sono le promesse che ci avete fatto l'anno scorso, l'estate scorsa, quando ci avevate detto che sarebbe stato tutto bello e che avremmo risolto tutti i problemi, andate in giro per le scuole italiane e vedete che cosa sta succedendo. Andate, ma non a farvi cantare le canzoncine dai bambini, come faceva Renzi: andate a vedere

che quanto sta accadendo quest'anno al sistema della didattica italiana andava messo in conto, però in buona sostanza il concorso per stabilizzare procede a rilento, i docenti di sostegno sono irreperibili, l'algoritmo ministeriale ha imperversato falcidiando sicurezze sociali

La seduta è tolta